la questione cioè della delega dei senatori a vita nell'ambito delle Commissioni, ovvero della delega di chi fa parte del Gruppo Misto e quindi ha uno*status*

estremamente variopinto. Signor Presidente, non voglio ridiscutere ora di questo problema, che spero venga ripreso dalla Giunta per il Regolamento, perché agli albori di questa legislatura la questione venne, secondo me, trattata in maniera sommaria. Oggi si è però verificato un episodio assolutamente paradossale: il senatore Cossiga, sostituito dal Capogruppo del Gruppo Misto con un altro collega, ha espresso tramite questo collega un voto favorevole sui presupposti di necessità ed urgenza relativi al decreto-legge sulla missione in Libano, quando è noto, diffuso, pubblicizzato e pubblicato che il senatore Cossiga era - e credo resti - contrario a tale missione. Il problema non è del senatore Cossiga, ma dell'istituzione Senato e del rispetto del ruolo, delle funzioni e delle caratteristiche proprie dei senatori a vita, e in particolare dei senatori che fanno parte del Gruppo Misto. Io sono ancora convinto

avrei voluto farle gli auguri di buon onomastico, ma non ho ancora capito se il suo nome è Franco o Francesco. Detto questo, vorrei collegarmi all'argomento introdotto dal presidente Pastore perché oggi la 1a Commissione ci offre molti argomenti. È accaduto - e vorrei che prima o poi qualcuno ci desse risposta

ha presentato una proposta di parere favorevole - non contrario - alla missione in Libano sull'esistenza dei requisiti di necessità ed urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione, motivandola come avvenuto in passato per le missioni di pace, citando un'espressione del presidente della Repubblica emerito Ciampi, che riunì sull'argomento il Consiglio supremo di difesa, quindi stiamo parlando non di un pericoloso esponente della Casa delle Dunque, presentiamo questa proposta di parere il Presidente della Commissione rifiuta di metterla in votazione perché sostiene che il parere favorevole va solo espresso, senza bisogno

Ora, se un parere contrario deve essere motivato, voglio immaginare che possa essere motivato anche un parere favorevole.

conclusione della vicenda è che a me e al collega Malan, per una certa coerenza che ci caratterizza evidentemente, si è sostanzialmente impedito di partecipare alla votazione, perché mi sono rifiutato di fronte a questo modo di procedere del Presidente della Commissione. Io credo che occorra ristabilire il diritto dei parlamentari non ad esprimere la propria opinione - perché questa non è una concessione che ci fa il Presidente di una Commissione - ma a proporre

Signor Presidente, prendo la parola perché credo sia opportuno lasciare a verbale qualche considerazione in risposta a quanto appena detto dai colleghi Pastore e Storace. Capisco che abbiamo avuto oggi in Commissione uno scontro piuttosto duro

a danno dell'opposizione da parte della maggioranza, né alcuna irregolarità. Questo, in particolare, per quanto riguarda l'operato del Presidente della Commissione e per quanto riguarda la maggioranza come soggetto politico che opera in Commissione. Come ha poc'anzi ricordato il collega Storace, ci siamo trovati a votare sui presupposti di costituzionalità di un decreto (in particolare, per conoscenza dell'Aula, il decreto sul Libano) e correttamente, secondo la prassi credo senza eccezioni seguita, il Presidente ha messo in votazione solo il sì o il no all'esistenza dei presupposti. È chiaro che ciascun collega dell'opposizione, in un contesto di questo genere, ha il diritto di motivare il suo sì o il suo no come vuole. Altra cosa è, però, avere un deliberato della Commissione che incorpora la motivazione, come avrebbero voluto i colleghi del centro-destra.

valutazione politica legittima, discussione politica legittima - e come abbiamo detto in Commissione, luogo appropriato per questa discussione certamente l'Aula del Senato ma non poteva questa valutazione, da parte loro legittima, che ci fosse una continuità tra le varie missioni all'estero essere parte di un deliberato della Commissione sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità di questo decreto, che era oggetto specifico del decidere della Commissione e che correttamente il Presidente della Commissione ha messo in votazione come tale. Mi pare evidente che le forze dell'opposizione, legittimamente, hanno cercato di provocare una difficoltà alla maggioranza; non è affatto censurabile e mi pare del tutto normale che questo accada, ma il luogo nel quale questo tentativo è stato esperito non era quello appropriato. Se lo vorranno, lo rifaranno! Sull'obiezione avanzata dal collega Pastore, vorrei che rimanesse a verbale in chiaro che i senatori a vita non sono senatori in parte diminuiti: sono senatori come tutti gli altri, che hanno funzioni e poteri eguali a tutti gli altri. Quanto Quanto alla sostituzione, dico con chiarezza soltanto che non siamo di fronte, Presidente, ad un mandato privatistico a rappresentare. Come ho detto in Commissione, questa non è un'assemblea di condominio, in cui io do il mandato come condomino ad essere rappresentato in un voto, espresso necessariamente dal mio incaricato in un senso o nell'altro, altrimenti viene meno al mio mandato. Questa è una sostituzione nella funzione politico-istituzionale: chi viene a sostituire ha diritto a tutto il rispetto e, soprattutto, ad essere riconosciuto nella pienezza dell'esercizio delle sue funzioni. di sostituirlo e mi dicesse: «Vai a votare così», gli risponderei: «No, grazie!» perché farei offesa alla mia autonomia ed indipendenza di parlamentare. Quindi, non si può rivolgere alcuna censura al voto che è stato legittimamente espresso in Commissione da parte di chi ha sostituito il senatore a vita. Riconosco poi la delicatezza del problema; anche qui c'è un punto sul quale, legittimamente, l'opposizione cerca di creare un problema alla maggioranza, ma secondo me poi la valutazione tecnica, giuridica, regolamentare e istituzionale della questione non deve prescindere da quelli che sono i parametri

a seguito di un confronto in Commissione vengono in Aula e sollevano la questione. Le pongo la questione, signor Presidente: in base a quale norma del Regolamento avviene una discussione di questo tipo? Se deve esserci una discussione, desidero poi che sia fatta in modo formale e che sia consentito al Presidente della Commissione e agli altri di poter intervenire per dire come si sono svolti realmente i fatti, poiché è stata offerta una rappresentazione dei fatti

Signor Presidente, dal 1982, quando è stata prevista nel Regolamento del Senato una deliberazione da parte della Commissione affari costituzionali circa la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza, mai, senza eccezione alcuna (anche quando Presidenti della Commissione erano colleghi autorevoli del centro-destra), è stata consentita come ammissibile la formulazione di un parere circa la sussistenza condizionato da valutazioni di carattere accessorio. cioè, o c'è o non c'è. Naturalmente nella motivazione della sussistenza dei requisiti i colleghi sono liberi di dire quello che ritengono opportuno dire. Analogamente a questa prassi, oggi non ho giudicato ammissibile la presentazione di un parere favorevole, ma nel quale era contenuta una valutazione accessoria, essendo ciò, ripeto, assolutamente difforme rispetto alla prassi. I colleghi hanno la possibilità - come hanno fatto - di motivare in sede di dichiarazione di voto.

dei requisiti di necessità e urgenza. Questa è prassi assolutamente costante e a questa ho inteso ispirarmi. Ciò nonostante, signor Presidente, ho ritenuto dal mio punto di vista opportuno investire della questione, per il futuro, la Giunta per il Regolamento e la Presidenza del Senato per dirmi se nel futuro si intende innovare rispetto a questa prassi e se ci sono valutazioni di questo tipo.

o meglio, il Presidente del Gruppo, che ha delegato altro senatore, il quale ha ritenuto di votare secondo quelle che sono le sue valutazioni. Credo che la valutazione sia politica e non di carattere procedurale.

del 7 giugno 2006, che ha lasciato un chiarimento di fondo. Comunque, quando in Aula viene posta la necessità di un approfondimento delle situazioni, non mi trincero dietro

Presidente, ovviamente non posso che apprezzare, condividere e sostenere le decisioni della Presidenza, cosa che farò comunque sempre. Però, poiché siamo ad inizio di legislatura e per cinque anni dobbiamo lavorare qui in Senato, vorrei rivolgerle una preghiera. Se ogni volta che i colleghi dell'opposizione hanno un problema, più o meno importante (non voglio giudicare), e questo viene considerato come un tema concernente l'ordine dei lavori, noi corriamo il rischio di parlare solo dell'ordine dei lavori. signor Presidente, vorrei chiederle la cortesia di essere un po' più rigoroso, perché altrimenti affrontiamo argomenti in Assemblea che con l'ordine dei lavori non c'entrano assolutamente niente. Capisco lo spirito, lo apprezzo e lo sostengo (oggi soprattutto si tratta di una questione di grandissimo rilievo); ma, signor Presidente, dovremmo anche cercare di tenere conto che la maggioranza ha l'interesse a procedere nelle votazioni. Senatore Boccia, la ringrazio. Non allunghiamo questo discorso, che avevo chiuso, per la verità. Ma, del resto, lei sui temperamenti non può influire. Io, quando si tratta di ascoltare, sull'ordine dei lavori, un'osservazione breve, com'è stata fatta dai senatori che sono intervenuti, ritengo che forse aiuti la gestione dei lavori di Assemblea nelle condizioni non semplicissime nelle quali siamo.

vorrei capire - e mi scuso se l'ha già detto e non sono riuscito a capirlo per la confusione che c'è - la sua risposta alla questione che le ho posto io, che è esattamente contraria a quella posta dal presidente Bianco.

reca il seguito della discussione Signor Presidente, ho chiesto la parola per pochi minuti perché ieri è scomparso Michelangelo Russo, che fu senatore dal 1992 al 1994. Fu componente di quest'Aula; ma, senza svalutare in nessun modo, ovviamente, questa altissima esperienza, che tutti condividiamo, vorrei ricordare molto brevemente Michelangelo Russo come dirigente politico, e come dirigente politico siciliano e grande meridionalista. Fu Presidente dell'Assemblea regionale siciliana in anni tragici per Palermo; erano gli anni dell'assassinio di Piersanti Mattarella ed erano insieme gli anni del compromesso storico. Io ricordo il suo legame personale di amicizia e di stima con Piersanti Mattarella ma ricordo anche che in quel rapporto c'era molto di più: più: la capacità di guardare alle questioni della politica siciliana, alle questioni della Sicilia e del Mezzogiorno con un'ambizione che oggi con difficoltà, colleghi - diciamolo guardandoci

E forse la ragione dei successi di quegli anni, la ragione anche del fatto che in quegli anni grandi figure politiche dominavano la scena siciliana e nazionale insieme a queste, quella di Michelangelo Russo, fu anche questa capacità di sfuggire alla tentazione di restare isolani a tutti i costi e di affrontare la questione meridionale con la cifra non della minorità, come spesso accade, ma, appunto, con l'attenzione di farne grande questione nazionale. Credo che in questo senso da quegli anni e da questi personaggi resti ancora viva per noi una lezione. Ho molti ricordi personali di Michelangelo Russo. Ho lavorato con lui, ho discusso con lui, ho litigato con lui. Abbiamo avuto momenti di disaccordo, ma questo mai ha potuto mettere in discussione la sua assorbente, totalizzante, autentica passione politica, la sua dedizione alla Sicilia e al meridionalismo. Negli ultimi anni ho lavorato nel suo centro studi e mi chiese più volte - scusate se mescolo questo ricordo personale al ricordo politico - notizie, informazioni, carte, documenti su temi stravaganti rispetto al suo impegno tradizionale: la tratta delle persone, il caporalato, la violenza sulle donne. Si poteva stupire solo chi non comprendeva il bisogno di un'intelligenza piena, cruda della realtà per cambiarla.

di chi pensa di essere simile agli dei e che per questa ragione non vuole cambiare niente, ma è anche la terra che ha espresso fattori straordinari e potenti di rivolgimento sociale, con le battaglie contadine e con la lezione ai contadini di non levarsi il cappello davanti al padrone. Michelangelo Russo era in questa tradizione politica, la tradizione politica che non ha paura delle proprie battaglie e della propria capacità di cambiare la realtà.

soltanto per dichiarare la disponibilità del Governo alla richiesta, avanzata dal presidente Salvi, di una breve pausa di sospensione.

La seduta è ripresa. Comunico all'Aula che il lavoro avviato con la sospensione di ieri è andato avanti, riconfermando l'intesa dei Capigruppo che questa sera si arrivi al voto finale sul disegno di legge in discussione anche, se necessario, con un breve allungamento dei tempi dell'Aula.

Con tutto rispetto della classe dei magistrati, credo bisognerà pure arrivare ad una soluzione. Se la soluzione comporta anche qualche ora in più, magari domani mattina, penso non sia un problema. Non lo dico in senso ostruzionistico:

per dare atto ancora una volta al Governo che sta compiendo grandi sforzi per arrivare ad una soluzione positiva e mi dispiace che in questo momento non sia supportato da tutta la sua maggioranza. Questo è un fatto politicamente significativo. Grazie,

che il Gruppo UDC si rimette alla sua saggezza: è al termine dell'ora di lavoro che sarà ragionevolmente comprensibile se occorre un'altra mezz'ora o no e confidiamo che la sua saggezza sarà tale da non impedirci l'accordo per mezz'ora, qualora fosse necessaria. Pertanto, ci rimettiamo alla sua saggezza in

Già nella riunione dei Capigruppo, che ha fissato il calendario per questo periodo, è stata indicata la chiusura per questa sera, con l'indicazione politica di arrivare alla conclusione dei lavori. Questo è avvenuto ed è stato comunicato

aggiornare, con l'intesa di tutti, la continuazione e la chiusura dei lavori per domani mattina. Il problema è legato proprio a tale impossibilità, che richiamo.

Speriamo che l'esito sia positivo. Come sapete, siamo stati fra i promotori di questo lavoro unitario. Mi rendo, quindi, anche conto delle esigenze che il presidente D'Onofrio e il presidente Castelli pongono. Credo sia possibile trovare un punto d'incontro, ma, come ci ricordava il presidente Marini, vi è

la sua richiesta, però vorremmo far presente un passaggio. Dato atto che si sta lavorando e che indubbiamente il lavoro è produttivo per tutti, teso a risolvere talune incomprensioni e quindi a costruire,

dati i tempi così stretti che lei propone, che ci troveremmo di fronte ad un cataclisma se questa sera entro le ore 21 non dovessimo votare il provvedimento. Lei sa benissimo, Presidente, anche per i fatti di ieri sera, che c'è stato un *vulnus* in questo provvedimento:

e non sulla graticola o tesi e strappati continuamente. Magari arrivati alle ore 19 non si sarà raggiunto nulla e forse si richiederà ancora tempo. Lo dico anche per la dignità dell'Aula:

senatrice Finocchiaro

Tra l'altro, vorrei ricordare ai colleghi due circostanze. La prima è quella sottolineata dal presidente Castelli, e cioè che stiamo ragionando su un testo che è stato oggetto dell'attenzione del Parlamento, in Commissione e in Aula, al Senato e alla Camera, per quattro anni e otto mesi e chi se ne è occupato, come i colleghi che stanno lavorando adesso, è totalmente padrone della materia. L'altra questione è che, se non dovessimo raggiungere l'accordo, ci resterebbero 14 votazioni da svolgere; e come pare sia assolutamente possibile, l'accordo si raggiungerà, avremmo soltanto un paio di votazioni da compiere e sarebbe inspiegabile che, avendo soltanto un paio di votazioni, l'Aula non venisse chiamata a votare e quindi ad alleggerire il lavoro complessivo del Senato da questo adempimento.

prego.

al Governo, in particolare ai sottosegretari Scotti e Maritati, e a tutti i membri della Commissione giustizia di entrambi gli schieramenti della serietà e dello spirito costruttivo con cui hanno affrontato questo difficile tema. Disponiamo ora di un testo che prevede la riforma della normativa sull'illecito disciplinare contenuta nella legge approvata nella passata legislatura. Con la stessa tecnica che si è seguita ieri per quanto riguarda l'altro decreto in questione,

che ora enuncerò in modo molto sommario e sintetico, ma se ci saranno richieste di chiarimenti questi potranno essere forniti. In primo luogo, si modificano le fattispecie di illecito disciplinare previste dalla legislazione vigente, nel senso di semplificare, ridurre ed eliminare quelle parti che ad alcuni potevano apparire compressive della dignità dei magistrati. Si è tenuto conto anche di alcune osservazioni - in particolare quella del presidente Andreotti, che non vedo - in merito alla riformulazione della disciplina che concerne i rapporti con i partiti e le forze politiche. Si è quindi proceduto ad una revisione delle fattispecie degli illeciti disciplinari, mantenendo il principio della tipizzazione, che è una grande novità che viene introdotta nel sistema perché, come i colleghi sanno, in questi ultimi sessant'anni non si era mai riusciti a varare una disciplina della tipicità degli illeciti disciplinari.

Si è però, come da più parti chiesto, introdotto un meccanismo di filtro, che consenta di esaminare preventivamente esposti manifestamente infondati o che concernono questioni a prima vista

Peraltro, come richiesto giustamente dall'opposizione, è previsto anche un meccanismo per evitare che questo filtro possa tradursi in realtà in rapide archiviazioni e così via. È pertanto prevista la possibilità di ricorrere contro la prima pronuncia di manifesta infondatezza, con un meccanismo che a nostro avviso garantisce sia l'esigenza di una certa rapidità del procedimento disciplinare sia quella del magistrato che fosse chiamato in causa di avere una chiara risposta, che quella del cittadino o di chi abbia proposto l'esposto di ricevere una risposta da parte dell'ordinamento. Si è infine eliminata la presenza - che è apparsa un duplicato di un delegato del Ministro in tutte le fasi del procedimento disciplinare e ciò per rispettare il sistema costituzionale, che al riguardo ha introdotto un sistema duale condizionato molto delicato che quindi va attuato in modo

Signor Presidente, ho letto l'emendamento 1.700, presentato dal relatore, e mi permetto di rappresentare al relatore stesso, per un'eventuale modifica, che in questo emendamento rimane fermo quel termine di un anno di decadenza, previsto per le varie scansioni di fase del procedimento disciplinare. Il ministro Mastella, nel suo intervento, aveva rappresentato come la ristrettezza di questo termine poteva, per certi versi, affaticare l'azione del Consiglio superiore della magistratura e principalmente, proprio in ragione tale ristrettezza, con riferimento all'aumento dei casi dovuti alla obbligatorietà dell'azione disciplinare, comportare una prescrizione continua degli illeciti disciplinari. Tutto ciò premesso, chiedo al relatore di voler valutare - se lo ritiene opportuno - di modificare il suo emendamento, nel senso di portare da uno a due anni il periodo di tempo concesso al procuratore generale per l'esaurimento della fase istruttoria e da uno a due anni il tempo previsto per la sezione disciplinare per l'emissione della relativa sentenza.

la partita delle occasioni perdute. Abbiamo potuto verificare che, laddove ci si è posti il problema di poter arrivare ad un accordo, ad un accordo si è addivenuti. Tuttavia, devo ricordare che in ogni caso l'articolo approva la sospensione - che in realtà, a mio parere, è una abrogazione - del decreto legislativo n. 160, che resta comunque assai importante. La separazione delle funzioni, l'accesso in carriera, la progressione in carriera vengono di fatto abrogate. Sono convinto che, se avessimo avuto più tempo, avremmo potuto affrontare positivamente anche questo aspetto; sono convinto che, se avessimo posto in essere l'atteggiamento che abbiamo posto in essere in questi giorni, anche durante i lavori in Commissione l'estate scorsa, oggi potremmo - credo con soddisfazione di tutti - votare a favore di un provvedimento che sarebbe stato a vantaggio non della sinistra, non della Casa delle Libertà, non dei magistrati, ma a vantaggio sicuramente di tutti i cittadini e della giustizia. Purtroppo,

vada avanti, senatore Colombo.

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, ero molto contento per il metodo con il quale si stabiliva un rapporto che non era manicheo né ostracistico degli uni o degli altri. Pensavo che questo - come ha detto benissimo il presidente Castelli - potesse essere, sia pure dal punto di vista della reminiscenza, un modo in cui procedere anche in altre occasioni. che sia stato giusto - com'è stato fatto opportunamente, ognuno dal proprio punto di vista, se è possibile - trovare convergenze su temi come quelliu concernenti la magistratura,

Si può discutere, semmai, di altro: accade, signor Presidente, che talune iniziative possano essere criticate e criticabili, e devono esserlo. Quando un potere, infatti, è senza responsabilità, si corre il rischio che diventi un prepotere e, forse, anche una prepotenza.

Per la prima volta dal 1993, con grande fatica e disponibilità intelligente di tutte le parti politiche (e rivendico, ancora una volta, il merito del mio Gruppo per aver cercato tale intesa fin dall'inizio), stiamo disancorando il sistema politico italiano dal blocco drammatico nel quale è caduto nel 1993. Stiamo cominciando una diversa navigazione, tutti insieme, anche nei confronti della magistratura, alla quale confermiamo rispetto e fiducia. Le due grandi novità che abbiamo introdotto sulla procura e sull'ordinamento disciplinare sono significative. Do per scontato che lo stesso faremo a proposito della separazione delle funzioni, ma è importante capire che in questo ramo del Parlamento italiano, per la prima volta dal 1993, si sta realizzando un significativo passaggio d'epoca. Per questo vorrei dire che non gradisco le dichiarazioni di guerra che ho ascoltato prima. *(Applausi

la volontà di voler alimentare in quest'Aula e fuori qualsiasi frizione. Gli incontri di oggi pomeriggio - i colleghi seduti al banco del Governo ne sono testimoni - hanno avuto anche momenti di significativa diversità di opinioni, all'interno dell'una e dell'altra coalizione, e mi hanno visto protagonista nel tentativo di non alimentare polemiche, anzi, nel limite del possibile, di sedarle.

dei cittadini, che hanno necessità di essere - loro sì - tutelati da coloro i quali, nell'ambito della loro stessa categoria, violano le regole e fanno perdere credibilità alla magistratura. Solo un processo equo ed effettivo dal punto di vista disciplinare può determinare questo. Signor Presidente, il senatore Furio Colombo, nelle ultime dieci ore, io non l'ho mica visto!

*(Commenti del senatore Castelli)*. No, presidente Castelli, non tenti di trascinarmi in una trappola o in una provocazione. Qualunque sia l'opinione dissenziente, da chiunque espressa in quest'Aula, non è un figuraccia. Vorrei dire a nome del mio Gruppo e mi permetta di dire anche a nome di tutti i colleghi dell'Unione - che il divieto di iscrizione ai partiti politici e l'eliminazione della possibilità di un conflitto di interessi con attività economiche o finanziarie, previsto da tale disposizione disciplinare, non solo è giustificata dal terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, non solo è prevista nel codice deontologico dei magistrati (per quanto riguarda il divieto di iscrizione ai partiti politici), ma risponde assai di più a un'esigenza costituzionale: quella che tutela l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, non come privilegio di una casta, ma come principio servente rispetto al pari trattamento di tutti i cittadini di fronte alla legge. Il dovere che l'Assemblea aveva nel legiferare su questo tema era esattamente quello di difendere il bene prezioso dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, ma guardandolo e interpretandolo come garanzia suprema dell'ordinamento per la parità di tutti i cittadini di fronte alla legge, nonostante le disparità di potere che li possono, nella società, contraddistinguere. Per questa ragione - come sapete - la nostra convinzione rispetto a questa parte dell'emendamento approvato

«*Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:* "Articolo 4-*bis*. Fino al 31 luglio 2007 continuano ad applicarsi, nelle materie oggetto del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, ed in particolare gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20. 2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e le situazioni esaurite durante la vigenza del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160"».

senatore Furio Colombo ha votato

vado avanti, ci mancherebbe altro! Non capisco, onestamente, per quale motivo si possa fare carico al senatore Furio Colombo, che ha votato con tutti noi l'emendamento della Commissione, di non aver partecipato ai lavori di una Commissione di cui non fa parte. Mi pare che abbia fatto benissimo a non venire.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,

Nella scorsa legislatura abbiamo - in quest'Aula - discusso molto di giustizia e molte leggi sono state emanate al riguardo. È vero, questo Paese ha urgente necessità di una riforma che renda il sistema giustizia più efficiente. La lentezza della nostra macchina giudiziaria non può essere disconosciuta. La possibilità di ottenere giustizia in tempi accettabili appartiene ancora, nel vissuto dei cittadini, a una mera ipotesi non suscettibile di concrete verifiche nella realtà. Tuttavia, nessuno dei provvedimenti varati nel corso della scorsa legislatura è riuscito a rendere la giustizia più rapida ed efficiente per le generalità dei cittadini.

Al contrario, sono state fatte varie leggi *ad personam* che hanno stravolto il funzionamento della giustizia. Un'assai controversa riforma varata nella XIV legislatura è stata proprio la riforma Castelli sull'ordinamento giudiziario. L*'iter* parlamentare di questa legge - come noi tutti sicuramente ricordiamo - è stato assai lungo e travagliato: dopo la sua prima approvazione definitiva nel dicembre del 2004, la «riforma» è stata rinviata alle Camere dall'allora presidente della Repubblica Ciampi per motivi di incostituzionalità. di incostituzionalità. Nel giugno del 2005 la legge è stata riapprovata con modificazioni dal Senato e nel luglio 2006 definitivamente dalla Camera. Pur ringraziando - in questo caso come SVP - la maggioranza di allora per la sensibilità dimostrata nei confronti dei problemi della giustizia nella Provincia autonoma di Bolzano, in special modo riguardo alla corte d'assise d'appello e al rispetto dell'impianto autonomistico, abbiamo sempre sostenuto che questa legge non soddisfa le esigenze di una giustizia equa e condivisa. Ma non intendo qui entrare nel merito della riforma Castelli e dei suoi effetti - a mio avviso - squilibranti dell'organizzazione giudiziaria. Intendo, tuttavia, evidenziare che la proposta del Governo in discussione, così come era stata approvata dal Consiglio dei Ministri ad inizio giugno, perseguiva lo scopo di evitare che al danno si aggiungesse la beffa. Perché, come illustrato nella relazione del disegno di legge governativo, la concreta operatività di alcune disposizioni della riforma Castelli comporta la tempestiva riorganizzazione di interi settori dell'apparato giudiziario. Per evitare un collasso del sistema giustizia che si sarebbe ripercosso, in definitiva, sui cittadini, il Gruppo Per le Autonomie aveva accolto con favore questo intervento del Governo che non intendeva abrogare la legge Castelli nel suo complesso, ma si limitava a disporre la sospensione di alcuni decreti legislativi attuativi della legge delega. Il provvedimento del Governo non si è mai ispirato a interessi di parte - un'accusa, lasciatemelo dire, strumentale e infondata - ma a esigenze di funzionalità della giustizia. Esso non va affatto visto come un colpo di mano, soprattutto perché è stato preannunciato a chiare lettere dall'Unione nel suo programma elettorale. Il centro-sinistra, infatti, aveva promesso che si sarebbe impegnato a rimuovere tutti gli aspetti del nuovo ordinamento in stridente contrasto con i princìpi costituzionali ed a intervenire con provvedimenti di sospensione dell'efficacia di quelle norme che potrebbero ledere il principio di unità, uguaglianza e parità di trattamento dei cittadini o le garanzie dell'indipendenza e autonomia della magistratura o rendere impossibile, successivamente, un nuovo e diverso riordino della magistratura. In ragione dei tempi richiesti per l'approvazione di un disegno di legge, sarebbe stata tuttavia più coerente da parte del Governo l'adozione di un decreto-legge di sospensione che avrebbe raggiunto lo scopo primario di questo provvedimento, ovvero impedire che i decreti legislativi attuativi della riforma Castelli divenissero efficaci alle scadenze per ciascuno di essi previste. Esprimiamo, tuttavia, soddisfazione per il fatto che si siano create successivamente le condizioni per un confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione sul disegno di legge in esame. A tal riguardo, uno speciale ringraziamento va soprattutto al ministro della giustizia Mastella, che in queste settimane si è fortemente impegnato per creare le basi per l'avvenuto dialogo tra i due poli.

Più complesso è stato invece trovare un'intesa sul decreto legislativo relativo ai procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. Anche su questo punto si è trovata, tuttavia, una soluzione ragionevole. stesso discorso vale per la questione delle carriere e della distinzione delle funzioni. Per trovare a tal riguardo un testo condiviso servono sicuramente tempi più lunghi. Per concludere, signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Per le Autonomie voterà a favore del provvedimento in esame per i succitati motivi e perché ritiene che l'approvazione di tale provvedimento ponga le giuste condizioni per continuare sulla strada già intrapresa di un riformismo serio. Serve, possibilmente in tempi brevi, una riforma il più condivisa possibile, che dia efficienza al sistema giustizia e insieme garantisca l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Tutto ciò non a servizio supino della magistratura, ma esclusivamente per attuare una giustizia davvero giusta per tutti i cittadini. *(Applausi

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi del Senato, il Gruppo Democrazia Cristiana-Partito Repubblicano Italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia esprimerà un voto contrario sul disegno di legge sulla sospensione dell'efficacia di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario. però evidenziare il lavoro proficuo che la Commissione e l'Aula hanno prodotto in queste settimane in un confronto serrato ma costruttivo fra posizioni inizialmente antitetiche che hanno trovato sintesi e punti di equilibrio accettabili per garantire il miglior funzionamento di un sistema delicato e complesso. E' questo un risultato della politica che ha la forza che gli deriva dal consenso democraticamente espresso dai cittadini. Perché se è vero che la Costituzione ha pienamente sancito il principio della separazione dei poteri e all'interno di questo sistema il ruolo primario del Parlamento, sede della sovranità popolare, è innegabile però che a partire soprattutto dai primi anni novanta, si è determinata nel nostro Paese una dialettica troppo aspra fra il potere giudiziario e la funzione legislativa del Parlamento. E' certamente un errore costruire una riforma dell'ordinamento giudiziario con il vizio di origine del conflitto con la magistratura, e questo non credo sia accaduto, ma è altrettanto sbagliato sospendere l'efficacia di tre decreti per adempiere ai desideri di qualche pezzo di magistratura militante. Oggi più che mai c'è bisogno di un rapporto fisiologico e di corretta dialettica istituzionale tra il ruolo del Parlamento e quello dell'ordine giudiziario perché abbiamo tutti la consapevolezza che il tema della separazione dei poteri non è pura simbologia della democrazia, ma garanzia di percorsi istituzionali in grado di affrontare in una corretta dialettica i bisogni dei cittadini. Siamo garantisti e non possiamo dimenticare alcuni eccessi che in questi anni si sono verificati nell'amministrazione della giustizia, quali l'uso distorto delle misure cautelari, la spettacolarizzazione dei processi, le invasioni di competenza ed una interpretazione talora ideologica della norma. Rispetto a questo noi riaffermiamo la necessità di assicurare l'uniformità dei criteri di esercizio della giurisdizione e quindi il principio della certezza del diritto e dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. A sostegno della necessità di sospendere l'efficacia dei decreti suddetti, veniva affermata dalla maggioranza, nella relazione introduttiva, la difficoltà di provvedere ad una tempestiva riorganizzazione di interi settori dell'apparato giudiziario. Sembrava questa una proposta irrinunciabile, una posizione pregiudiziale, un punto politico di discontinuità e contrapposizione. Le Assemblee legislative, attraverso i loro atti, segnano i tempi, codificano il pensiero comune, le convinzioni collettive, accompagnano la crescita di comportamenti, valori e tendenze. Questo bipolarismo muscolare e forzoso invece crea il convincimento che ogni volta che il Governo del Paese cambia, si debbano riscrivere per intero le norme espresse dalla maggioranza precedente, in maniera alternativa, senza impegnarsi invece in un lavoro di perfezionamento sulla base delle esperienze maturate. Laddove la contrapposizione politica è così accesa, come sul terreno dell'ordinamento giudiziario, la tentazione è quella di abrogare *tout court* il lavoro precedente per segnare una discontinuità. La sospensione dell'efficacia dei decreti nn. 106, 109 e 160 sarebbe andata in questa direzione ma, come dicevo prima, le leggi devono esprimere le convinzioni, i valori e gli interessi del Paese. Le esigenze del Paese in buona parte si rintracciano nei tre decreti Castelli. Che questo sia vero lo dimostrano le perplessità di ampi settori della maggioranza e l'*iter* parlamentare dei provvedimenti. Infatti, questa Assemblea ha dato una risposta per molti versi equilibrata e lungimirante ai problemi posti. Le modifiche minime al decreto n. 106, in cui si postula «assegnazione» e non la semplice «delega» ai sostituti, garantisce insieme l'autonomia dei sostituti e consolida il ruolo di indirizzo e di garanzia del procuratore capo. La mediazione così raggiunta ci pare salvaguardi la sostanza del decreto Castelli. Possiamo certamente dire che questo risultato è frutto della compattezza dell'opposizione in quest'Aula ma anche dell'attenzione alle nostre ragioni di alcuni settori della maggioranza. Voglio sottolineare per tutti l'intervento del collega Di Lello Finuoli che ha aperto uno spazio per la riflessione nella maggioranza e soprattutto l'attenzione del Ministro, che ha dato prova di pragmatismo, flessibilità, e capacità di mediazione. Ascoltare, comprendere le ragioni di tutti, decidere per i bisogni reali dei cittadini è il compito dei parlamentari. Verremmo meno ad un obbligo della democrazia se ci trasformassimo in portavoci faziosi di gruppi di potere o di pressione o peggio ancora di quanti operano per una delegittimazione del Parlamento. D'altra parte, anche il voto di ieri dell'Aula, che ha visto anche la maggioranza sconfitta, conferma il prevalere delle ragioni della dialettica parlamentare su ogni posizione pregiudiziale. La maggioranza è certamente venuta meno per un suo problema interno, marcata com'è da elementi di debolezza strutturale, ma anche per la complessità delle posizioni che si sono palesate in questo campo così delicato e difficile. Siamo consapevoli, per esempio, che sul tema della distinzione delle funzioni tra magistratura giudicante e magistratura inquirente vi è una disponibilità vera al merito del confronto, per costruire una soluzione di garanzia in linea con quanto avviene negli ordinamenti di altre grandi democrazie occidentali. Ma, allo stesso tempo, non si può limitare il giudizio sul decreto n. 160 alla postulata separazione delle carriere, dimenticando l'obiettivo, che il decreto si pone, di migliorare il sistema di accesso alla magistratura per una maggiore professionalità e indipendenza dei futuri magistrati. Anche oggi, per quanto riguarda il decreto n. 109, la Commissione giustizia ha lavorato per individuare una soluzione che rappresenti un auspicato equilibrio tra i princìpi di responsabilità, che devono caratterizzare l'attività dei magistrati, e le esigenze di garanzia, che derivano dalla tipizzazione delle condotte censurabili sotto il profilo disciplinare. Il confronto, qualche volta duro, di questo decennio tra il potere legislativo e l'ordine giudiziario, la tentazione di alcuni partiti di schierare al proprio fianco la magistratura e di farsene garante politico, hanno determinato un clima inaccettabile relativamente ai temi dell'amministrazione della giustizia nel nostro Paese, facendo dimenticare le questioni reali e producendo un grave disorientamento dei cittadini.

C'è un convitato di pietra in quella che sembra una partita a due tra politici e magistrati: il cittadino che attende troppo a lungo o inutilmente una giustizia giusta, il cittadino che chiede professionalità dai magistrati e certezza del diritto. Con questo obiettivo, colleghi, vanno valutate le norme relative all'accesso in magistratura e alla formazione culturale e permanente dei magistrati e va considerata, nella logica di una corretta dialettica processuale, la distinzione certa tra funzione inquirente e funzione giudicante. Certamente oggi i cittadini non possono dirsi soddisfatti di questo livello dell'amministrazione della giustizia e questo per responsabilità diffuse. I tre «decreti legislativi Castelli» - li chiamo così per semplificare - si ponevano quale tentativo serio di dare risposte efficaci a queste necessità. La maggioranza, secondo una corretta logica parlamentare e politica, avrebbe dovuto presentare una proposta migliorativa, un suo progetto complessivo, e non solo una sospensione cautelare. Ma questo avrebbe richiesto una forza e una consapevolezza delle proprie ragioni che questa maggioranza oggi non possiede. Da ciò l'esigenza di sospendere oggi, e forse sopprimere domani, l'efficacia dei decreti Castelli. Il percorso parlamentare ha consentito, invece, di liberarci e liberare il Paese, almeno in questo caso e solo parzialmente, da questa camicia di forza degli schieramenti, approdando a soluzioni in qualche modo condivise. I dubbi, i ripensamenti, le sintesi di mediazione raggiunti non sono frutti casuali, ma dialettica parlamentare, il sale della democrazia, il prevalere, quindi, del buon senso e dell'interesse generale sulle posizioni pregiudiziali che ha fatto da argine, almeno per una volta, a questa vocazione diffusa, autodistruttiva, della militarizzazione della politica. Per questo, il voto contrario che il nostro Gruppo esprime sul complesso del provvedimento in discussione in questa occasione ha un contenuto e sfumature del tutto diverse dalle altre questioni finora trattate in quest'Aula.

Presidente, onorevole Ministro, il Gruppo dell'UDC vota su questo provvedimento, originariamente proposto dal Governo, con qualche difficoltà. Noi capiamo che votiamo contro un provvedimento alla radicale modifica del quale abbiamo concorso in modo decisivo. Se avessimo voluto far precedere le ragioni del metodo seguito nella modifica del provvedimento alle ragioni del fatto che quest'ultimo venga dal Governo, avremmo dovuto votare a favore di questo provvedimento. Noi votiamo contro perché, ovviamente, si tratta di un provvedimento che, sebbene ridotto ad un terzo soltanto della disposizione iniziale (che riguardava procure della Repubblica e procedimento disciplinare), è pur sempre un provvedimento che prevede la sospensione di un decreto di un decreto legislativo attuativo di una riforma voluta da questa parte politica, che era maggioranza nella precedente legislatura. Ho detto prima e ripeto ora che il nostro voto contrario è sostanzialmente un voto che parte dalla constatazione

Per una ragione politica molto importante: questo provvedimento è giunto al Senato con la caratteristica della sospensione di fatto dell'intera riforma dell'ordinamento giudiziario approvata dal centro-destra nella precedente legislatura. A questa ipotesi noi abbiamo contrapposto con forza, con tenacia, con una capacità di iniziativa che pochi credevano possibile, l'ipotesi che in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario non si potesse procedere più con l'idea che una maggioranza può fare quello che vuole, ma che, trattandosi di regole istituzionali, si dovesse cercare dovunque l'intesa per una riforma stabile, qualunque parte politica vinca le elezioni. Ritengo che, da questo punto di vista, il comportamento del Governo e della maggioranza che lo sostiene, nonostante le difficoltà procedurali alle quali abbiamo assistito, nel corso di questi tre mesi sia cambiato anche per merito nostro. Rivendico con forza il merito dell'UDC per aver detto, fin dal luglio scorso, non nelle ultime ventiquattro ore, che su questa materia era necessario capire se il Governo voleva abrogare o modificare la riforma Castelli. La proposta un po' furbesca di sospendere il provvedimento Castelli di fatto poteva diventarne l'abrogazione, se la sospensione fosse stata caratterizzata da una volontà di chiudersi, come maggioranza, a riccio. Ciò non è avvenuto. Abbiamo posto una sfida, signor Presidente; abbiamo posto una sfida, signor Ministro. Volevamo capire se, sulla materia dell'ordinamento giudiziario, le due caratteristiche di fondo della proposta Castelli Castelli (il potere esclusivo del procuratore capo della Repubblica nell'inizio dell'azione penale e l'obbligatorietà dell'azione disciplinare), quei due pilastri rimanevano intatti o no. Ci è stato detto che questi pilastri rimangono, con le modifiche che hanno ritenuto giusto apportare ad essi. Abbiamo detto, a questo punto, che è ovvio che procura della Repubblica e procedimento disciplinare saranno diversi da quelli della riforma Castelli, che non viene quindi abrogata, non viene più neanche sospesa, ma viene modificata, come ritenevamo doveroso. È per queste ragioni che noi riteniamo che anche la terza parte della riforma Castelli, quella corposa, che riguarda la separazione delle funzioni, di fatto poteva essere modificata d'intesa all'inizio di questa legislatura, senza alcuna sospensione del del decreto legislativo n. 160 del 2006 dell'allora ministro Castelli. Ciò non è stato possibile. Ma è evidente che il voto finale su questo disegno di legge - è bene che i colleghi della maggioranza colgano questo punto - non è più il il voto a favore di un disegno di legge che comportava di fatto una sospensione generalizzata del provvedimento; è diventata residuale. Noi riteniamo che, da questo punto di vista, l'introduzione della separazione delle funzioni dovrà tenere conto, in misura notevole, del fatto che le procure della Repubblica sono caratterizzate dal potere esclusivo (che il disegno di legge mantiene) dell'azione penale da parte del procuratore capo e dall'obbligatorietà dell'azione disciplinare. Ecco perché il nostro voto è, in un certo senso, contrario per ragioni formali e procedurali, è politicamente un voto favorevole. Noi cogliamo nella ragione dell'intesa sulla riforma dell'ordinamento giudiziario un punto strategico al quale più volte il Ministro si è richiamato nei suoi interventi, nei suoi interventi, ai quali mi sono riferito più volte negli interventi a nome del Gruppo UDC, e che abbiamo visto con grande soddisfazione diventare anche oggi, quando sembrava imminente la rottura definitiva tra le due parti politiche. Abbiamo detto che era soltanto un intervallo procedurale e politico, non era una conclusione negativa. L'altro ieri, quando sembrava definitivamente conclusa in modo negativo l'intesa sulla riforma delle procure, abbiamo detto che c'era un supplemento di intesa possibile. Quando il ministro Mastella ha chiesto di accantonare senatore Caruso su questo argomento, abbiamo dato la disponibilità, perché abbiamo capito che nella richiesta di accantonamento del Ministro non vi era solo una ragione di compattezza della maggioranza che sostiene il Governo, ma vi era anche una ovvia disponibilità a capire se le ragioni che noi avevamo indicato erano componibili con le ragioni della maggioranza. In questo senso credo abbia ragione la collega Finocchiaro quando parla di una vittoria del Parlamento.

di svincolarsi dal proprio schieramento per chissà quali intendimenti politici. Vi era soltanto l'intendimento serio, questo sì, di passare dalla logica dello scontro militarizzato dei blocchi contrapposti alla ricerca dell'intesa sulle regole istituzionali. Noi continueremo lungo questa strada, dando per scontato che la maggioranza che sostiene il Governo e il Governo stesso cercheranno l'intesa anche sulla questione della separazione delle funzioni e, una volta che tale intesa sarà raggiunta, non avremo difficoltà ad esprimere un voto favorevole, come abbiamo fatto in merito alla riforma della

la soluzione del problema,

i quali separatamente lasceranno a verbale le proprie dichiarazioni di voto, L'esposizione sintetica del presidente Salvi mi esime dal tornare sugli aspetti qualificanti

che se volessimo, come maggioranza, emettere un bollettino di vittoria dovremmo anche ricordare la buona volontà dell'opposizione con la quale in due o tre giorni di trattative, pur rimanendo ognuno nell'ambito delle proprie convinzioni, abbiamo trovato un accordo che che può essere un segnale non tanto ai magistrati quanto ai cittadini.

Una riforma condivisa dà forza, non solo all'ordinamento giudiziario, ma anche al sistema giustizia. E quel che oggi manca in Italia è

È vero, è una vittoria del Parlamento, ma è anche una vittoria dei cittadini, i quali, specialmente sul disciplinare, oggi sapranno essere tutelati. I magistrati invocavano da anni una tipicizzazione degli illeciti disciplinari. Noi l'abbiamo ottenuta sfrondando la legge Castelli da tutte quelle forme vaghe di chiusura che portavano la tipicizzazione ad essere vanificata. Abbiamo invece, con la buona volontà dell'opposizione, trovato delle forme di tipicizzazione

Abbiamo quindi tutelato con questa riforma anche i cittadini, che sono i primi beneficiari di un sistema giudiziario serio e condiviso. L'indipendenza della magistratura è sempre stata il faro delle nostre riflessioni e delle nostre battaglie. Credo che con questa riforma del disciplinare il sistema della protezione dell'indipendenza della magistratura venga rafforzato, perché il magistrato non sarà in balia del Ministro o del procuratore generale della Cassazione in base a dei comportamenti che magari a Milano vengono tollerati e a Bari no. Oggi ci sarà un'uniformità di riferimento dei comportamenti, insieme, ovviamente, all'obbligatorietà dell'azione disciplinare, perché sarebbe stato

non dovremo farci coinvolgere da ideologismi, bensì guardarci intorno in Europa. L'ho detto anche all'inizio di questa discussione: la divisione delle carriere non può essere un tabù, perché è prevista in tutti i Paesi europei. In Italia possiamo comunque raggiungere un buon accordo sulla divisione delle funzioni,

Queste sono le assicurazioni che come maggioranza possiamo dare. Non siamo per l'abrogazione di questa importante parte della riforma. Non siamo per scatenare guerre religiose, ma per andare avanti, ognuno nella chiarezza delle proprie posizioni e nella fermezza dei propri princìpi. Vogliamo andare avanti per riformare veramente la giustizia italiana. Credo che il mio intervento, svolto a nome di tutti i partiti dell'Unione, possa dimostrare

Signor Presidente, colleghi, credo che prima di tutto occorra fare alcune considerazioni di natura politica su questa vicenda, che, come ho ricordato prima, dura ormai da quasi cinque anni, a dimostrazione incontrovertibile di come sia stato faticoso e difficile legiferare su tale materia. La prima considerazione che si può fare è che il Parlamento,

incontrovertibile: è il Parlamento che fa le leggi, tutti gli altri soggetti vi si devono adeguare. La seconda considerazione che possiamo fare riguarda un dato di fatto: finalmente la verità è venuta a galla. Ricordo gli insulti, le polemiche, le affermazioni apocalittiche secondo le quali anche soltanto un minuto di vigenza della riforma dell'ordinamento giudiziario introdotta dalla Casa delle Libertà

legislativo più controverso, il n. 160 del 2006, probabilmente verrà ad esplicare per qualche mese o per qualche giorno i suoi effetti. Ma lasciamolo pure da parte:

e moltissimi parlamentari che oggi siedono in questo Senato hanno partecipato a questa grande fatica - deve sentirsi orgoglioso, perché ha consentito al Paese di fare un passo in avanti. Mi riferisco a quanto diceva prima il senatore Andreotti, e cioè che addirittura neanche la Costituzione stessa è riuscita a dire una parola definitiva sull'attività politica dei magistrati; noi ci siamo riusciti e abbiamo dato un quadro preciso, definitivo e, credo, soddisfacente per tutti. Da un lato, viene salvata Da un lato, viene salvata l'incontrovertibile prerogativa costituzionale per la quale il magistrato, da cittadino, può esprimere le proprie idee, ma viene anche statuito che il magistrato non è un cittadino qualunque; ha guarentigie, diritti particolari e quindi anche doveri particolari di correttezza, equidistanza e pertanto non può partecipare direttamente all'agone politico. Altro non fosse se non per questa norma, noi avremmo fatto un lavoro positivo. Ve ne moltissime altre; non ritorno sulla questione dell'ufficio del procuratore che credo sia veramente una svolta epocale; finalmente dà ordine in un'attività così delicata, così fondamentale

perché si era instaurato un clima di collaborazione; sarebbe stato bello e positivo poter coronare questo clima con una luce verde. Non ci è consentito perché c'è stata una mancanza di coraggio da parte della maggioranza; non si è osato affrontare l'ultimo *totem*, l'ultimo tabù: la separazione delle funzioni, ma soprattutto la meritocrazia nella progressione in carriera dei magistrati. Bisogna pure affrontare questo tema, colleghi. Chi di noi stasera non è qui per merito? C'è qualcuno di noi che forse stasera non è qui per merito? Non credo. Ciascuno di noi ha una storia personale dietro che, attraverso una serie di impegni personali, di studio, di applicazione, del fatto che ci si è messi in gioco, ci ha consentito di arrivare in quest'Aula. Chi delle persone che fuori lavorano non progredisce, non va avanti nella vita per merito? Nessuno. Bene, abbiamo una sola categoria che è avulsa da questa logica scontata per tutti: è la classe dei magistrati. Credo che su questo tema dovremo pur confrontarci; non si è avuto il coraggio di farlo ora - secondo me è un peccato -, non si è avuto il coraggio di affrontare il problema della separazione delle funzioni; lo si poteva fare perché in via privata, molti, anche esponenti dell'attuale maggioranza, mi hanno confessato che il primo testo che avevamo presentato al Senato era un testo che poteva essere assolutamente praticabile e affrontabile. Consentitemi una nota pessimistica: non credo che potremo tornare tanto facilmente su questi temi in questa legislatura, anche per una questione pratica. Ho ricordato prima come abbiamo passato ore e ore a discutere; anche questa legislatura ha impegnato ha impegnato l'Assemblea quasi totalmente su questo tema. È chiaro che il Paese aspetta anche la risoluzione di molti altri problemi, altrettanto e forse anche più gravi. Questo Questo era il treno che avremmo dovuto prendere; lo abbiamo perduto e non so quando tornerà. Questo è il motivo che ci costringe a votare contro.

siamo al momento del riassunto dei nostri lavori e quindi riassumiamo. Il Ministro si è affacciato nell'Aula del Senato con questo disegno di legge con cui ha proposto di sospendere tre decreti legislativi attuativi della riforma dell'ordinamento giudiziario voluta e votata dalla maggioranza di centro-destra nella XIV legislatura, più un altro intervento di non poco conto. Il Ministro si è affacciato in quest'Aula con un disegno preciso: colpire al cuore la riforma dell'ordinamento giudiziario voluta e votata dalla maggioranza di centro-destra nella XIV legislatura. Il Ministro esce da quest'Aula con due dei tre decreti legislativi modificati marginalmente, in maniera infinitesimale (con riferimento al principale, quello che riguarda

saranno felici di questo risultato, che oggi il Ministro guardasigilli e la maggioranza di centro-sinistra ottengono: può darsi di sì, può darsi di no. Nel caso in cui siano felici, è ovvio che la felicità sarà quantomeno mitigata dal fatto che - è notizia di oggi - l'articolo 65 del disegno di legge finanziaria voluta dal Governo di centro-sinistra un qualche dispiacere loro lo dà, diminuendone gli emolumenti

all'indipendenza e all'autonomia della magistratura. Insomma, un attentato che va ed uno che viene. Quello che va, purtroppo, è quello che doveva essere recato dal decreto delegato sul riassetto delle carriere

Il ministro Mastella esce dall'Aula senza avere più l'articolo 3, che era un altro colpo al cuore - e non da poco - all'operazione trasparenza che il Gruppo di Alleanza Nazionale - devo

alla quale il ministro Mastella aveva cercato di inferire un colpo al cuore, e che, viceversa, è restata e resta nel nostro ordinamento.

La sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo che rimane (quindi quello sul riassetto delle carriere), tuttavia sospende, azzera e quindi inferisce un vero colpo al cuore al principio della separazione delle funzioni, che rappresentava il contenuto più innovativo e davvero di svolta della riforma dell'ordinamento giudiziario da noi voluta.

sulla circostanza che i magistrati eletti, gli avvocati e i docenti universitari designati non fossero all'altezza di interpretare ed attuare la riforma dell'ordinamento giudiziario, ma avessero bisogno di un periodo di tirocinio, è semplicemente offensivo per costoro. Ma è offensivo anche per l'intelligenza del Parlamento, perché quando si vuole sospendere e basta significa che non si sa cosa si vuole fare, significa un'assoluta confusione sul programma della giustizia. Badi, signor Ministro, non so cosa sia successo dopo. Lei è corso ai ripari, ma intempestivamente, perché nelle dichiarazioni programmatiche del Governo in Commissione giustizia non ha detto nulla, e d'altra parte molti esponenti dell'Esecutivo e della maggioranza sostenevano che sarebbe stato il Parlamento poi a rivisitare la riforma dell'ordinamento giudiziario. Lei è corso ai ripari (ci fa piacere) con una serie di dichiarazioni programmatiche estremamente generiche, di cui non abbiamo ancora visto l'attuazione in concreto e che possono prestarsi anche a modifiche assolutamente destabilizzanti rispetto all'*incipit* principale.

con un confronto assolutamente onesto, leale e serrato tra maggioranza e minoranza, di arrivare ad una sintesi veramente soddisfacente per tutti ma, soprattutto, che ha condotto a una vittoria contro gli estremisti della politica. fine, infatti, ci si rende conto che gli impianti dei decreti delegati sulla procura e sulla materia disciplinare tanto demonizzati, che in campagna elettorale erano stati sbandierati come momenti di assoluto ripudio da parte dell'Unione, andavano bene,

Hanno funzionato e alla fine sono stati modificati solo in misura assolutamente marginale. Il decreto delegato sulle procure vede rafforzata la figura del procuratore della Repubblica come titolare esclusivo dell'azione penale, quale può assegnare un procedimento al sostituto, ma glielo può togliere, se non risponde ai criteri che gli ha indicato, senza che vi sia nessun organismo a cui rivolgersi. il portavoce per i *media* dell'ufficio, che eviterà quei protagonismi e quei rapporti patologici dei magistrati con i mezzi di comunicazione che tante devastazioni e tanti problemi hanno provocato per i diritti fondamentali dei cittadini. Lo stesso procedimento disciplinare è stato modificato solo in parte. Diceva bene il collega Castelli: abbiamo avuto il coraggio di toccare dei punti sensibili.

abbiamo sancito il divieto di partecipazione sistematica e continuativa, seppure in modo informale, ai partiti politici, cosa che molti magistrati hanno l'abitudine di fare.

se il decreto-legge Biondi non fosse stato ritirato dal Governo. Un vero e proprio colpo di Stato, che si voleva porre in essere da parte della magistratura militante e politicizzata. Abbiamo regolato i rapporti con la stampa e con la politica, punti fondanti per affermare una vera autonomia e una vera indipendenza della magistratura. Con queste norme vincono i magistrati, quelli che svolgono il proprio dovere, in silenzio, lavorando, rischiando la vita e pagando con la vita.

Perdono coloro che, forti di una posizione politicamente rilevante, in uscita dal Consiglio superiore della magistratura avevano magistratura avevano l'abitudine di scegliersi i posti da ricoprire successivamente. Una funzione così alta, come quella del Consiglio superiore della magistratura, non può assolutamente essere sporcata con questi comportamenti da bassa bottega

però fermati al punto fondamentale, signor Ministro: la separazione delle funzioni, i concorsi. Ho apprezzato le sue dichiarazioni, nel senso di prevedere la distinzione delle funzioni: vedremo come. Ho apprezzato anche le dichiarazioni del collega Di Lello Finuoli in merito ad una separazione delle funzioni, che non rappresenta più un tabù assolutamente intoccabile. Non so se poi tutto ciò ve lo faranno attuare, se poi, in concreto, tutto ciò verrà attuato. Ed è stato un peccato, perché se avessimo cominciato da subito a discutere nel merito e non solo di sospensione, oggi probabilmente

sul programma giustizia, non solo sulla separazione delle funzioni, che è un punto fondante. Che fine ha fatto la riforma del diritto penale? Vi sono state due Commissioni nella XIII e nella XIV legislatura che hanno lavorato. Che fine ha fatto questa riforma? Che fine ha fatto la riforma del processo penale, voluta da tutti e che ha visto nella XIII legislatura una serie di riforme coerenti e logiche, come quella dell'articolo 111 della Costituzione, e assolutamente illogiche e incoerenti, come quelle della cosiddetta legge Carotti?

Sono veramente curioso di sapere se, dopo tutte queste misure negative rispetto alle richieste dell'ANM, verrà meno il silenzio assordante di coloro che ieri, con bilanci inalterati del Ministero della giustizia e anzi aumentati, con una serie di riforme utili ai magistrati e alla loro attività, strillavano come aquile per la mancanza della carta. Certo, dopo i tagli del decreto Bersani

Oggi ha vinto la magistratura e sono stati sconfitti i magistrati militanti e politicanti. *(Applausi dal Gruppo FI).* Spero che domani avvenga lo stesso, ma soprattutto è importante che continui a vincere la politica, nell'accezione alta del termine, scevra da condizionamenti esterni. Una politica che tenda ad un quadro di sistema e non certamente ad una popolarità a ogni costo. Una politica dotata di una visione coerente, omogenea. Signor Ministro, la politica del centro-sinistra è frammentata, è ostaggio di estremismi, vive di agguati, è semplicemente incoerente. In una parola, signor Ministro, non solo sul sistema giustizia, ma su tutto il sistema Italia, voi siete incapaci di governare questo Paese e di farlo progredire.

e vorrei, in conclusione, ringraziare innanzitutto la mia maggioranza che mi ha sostenuto e anche quelli al suo interno che hanno avuto qualche perplessità, qualche dubbio o qualche reticenza;

Non c'erano legionari o crociate da mettere in moto rispetto ad altri poteri e rappresentazioni istituzionali autonome della vita del nostro Paese.

e quanti hanno collaborato alla stesura finale. Credo che questa sia una buona occasione per tutti e ringrazio davvero in maniera eguale tutte le parti e tutti gli appezzamenti del territorio parlamentare.

sentirlo? Il titolo è: «Sospensione dell'efficacia» - tanto per cominciare - «nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario». il seguente:* «Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario»